Signor Presidente, intendo rimettermi alla relazione scritta. Per ulteriori informazioni di sintesi ai colleghi, Convenzione risale all'epoca del precedente Governo; da qui probabilmente la comprensibile sollecitazione di tutti i colleghi del Partito Democratico,

non sempre facilmente prevedibili rispetto ai nostri calendari di Aula, direi che essi sono stati abbastanza solleciti.

vincolante per i diritti, le dignità, le pari opportunità riconosciute alle persone con qualsiasi tipo di disabilità. Essa si riferisce a tutti gli aspetti della tutela e della promozione delle persone con disabilità, che sono considerati ovviamente all'interno della tutela dei diritti umani; mi riferisco al diritto alla vita, all'integrità fisica, alla tutela giuridica, alla sicurezza, alla protezione sociale, all'istruzione.

nella sua interezza, vediamo che invece molto spesso vengono calpestati, talvolta neppure riconosciuti. È un provvedimento per il quale gli Stati si impegnano ad assicurare un sistema inclusivo a tutti i livelli, l'apprendimento a lungo termine, garantendo che le persone con disabilità non siano escluse dal sistema educativo generale e che i bambini disabili siano integrati nella scuola gratuita ed obbligatoria. È poi riconosciuto un ruolo importante e fondamentale alla famiglia, intesa come gruppo sociale di base, deputata a proteggere le persone con disabilità.

è frutto di un percorso partecipato, in quanto i lavori preparatori hanno visto un ampio coinvolgimento della società civile. Come tutti i processi partecipati, il frutto ha una particolare importanza perché in qualche modo ci garantisce una applicazione applicazione delle norme in esso contenute più facile, proprio perché condivise. Il testo del documento è stato negoziato ed elaborato con ampie rappresentanze anche delle associazioni per i disabili, le quali si sono fatte portatrici delle istanze concrete che questo mondo richiede e di cui ha bisogno. La Convenzione poi individua, quali azioni fondamentali, la lotta ad ogni forma di discriminazione dei disabili e la promozione dell'uguaglianza e delle pari opportunità.

La Convenzione vieta qualsiasi forma di discriminazione e impegna le Nazioni che l'hanno sottoscritta, e che compongono l'Assemblea generale, ad adottare leggi che proibiscano discriminazioni basate su qualsiasi forma di disabilità, dalla cecità alla malattia mentale. cari colleghi, la Convenzione dedica una particolare attenzione ai bambini disabili, un fatto a mio avviso molto importante.

è previsto espressamente il diritto alla vita e si impegnano gli Stati a mettere in atto misure perché questo accada. Mi sarebbe piaciuto che anche il Vaticano, oltre ad avere contribuito a redigere il testo della Convenzione, avesse potuto sottoscriverlo, perché quello dei diritti e, soprattutto, dei diritti delle persone con disabilità è un tema troppo importante a cui nessuno credo possa sottrarsi nell'attenzione e nell'adozione di misure che ne consentano la tutela. *(Applausi dai Gruppi

quindi, di sostituirmi al relatore, nel ricordare alcuni dei punti fondamentali che vengono elencati all'articolo 3 di questa Convenzione. Si dignità, autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, non discriminazione, piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società, rispetto delle differenze delle persone con disabilità, pari opportunità, accessibilità, parità di genere e rispetto per lo sviluppo e per l'identità dei bambini con disabilità, com'è stato ricordato questi aspetti si stabiliscono non solo nuovi diritti per persone con determinati problemi (la Convenzione elenca quali siano da ritenere le disabilità al centro di questo

Che cosa si intende fare con questo documento? Si intendono abolire tutte quelle barriere che non consentono l'agire civile, politico, economico, sociale - e quindi anche culturale di milioni e milioni di persone. Persone che in questi anni sono state tenute nel silenzio non soltanto da una serie di politiche che le hanno escluse dalla partecipazione attiva alla società, ma anche, com'è stato ricordato, da ricordato, da tutta una serie di comportamenti di tipo paternalistico, che includevano i disabili in una categoria indefinita di malati, verso i quali ci si doveva comportare in maniera commiserevole, senza mai riconoscere loro il benché minimo diritto. Questa Convenzione dovrà poi essere non soltanto ratificata, ma anche inclusa nel nostro ordinamento. Per far ciò, non solo dovrà essere creato un organismo che viene chiamato Osservatorio, ma dovranno altresì essere trovati fondi per poter finanziare

Ho avuto modo di essere presente non soltanto alla fase finale dei negoziati - quando rappresentavo il Partito Radicale transnazionale alle Nazioni Unite - ma anche quando il ministro Maroni, due legislature fa, ritirò

rassegna delle nostre leggi. Ora, sappiamo che in Italia tra le leggi, le politiche e l'effettivo godimento dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali vi è spesso, se non un oceano, sicuramente un mare. Ecco, questo mare, da quando

consegnati all'allora ministro Maroni, ma non si è trovato il modo di adottare una serie di misure che avrebbero dovuto iniziare ad abbattere le barriere che ancora separano i disabili dal pieno godimento dei diritti di cittadinanza. Quindi la ratifica che ci apprestiamo a votare quest'oggi, che vede tutti noi favorevoli, nello spirito e nella lettera della Convenzione - forse un po' meno della legge di ratifica - dovrà dare il "la" ad una serie di stanziamenti finanziari relativi a misure che intendono in qualche modo recuperare il tempo perduto e, finalmente, riempire di fatti

dei disabili. Ebbene, nessuna misura è stata ancora presa perché i disabili intrasportabili ed i malati gravi possano votare in occasione delle elezioni. Si tratta di una riforma che, secondo stime

oltre che garantire, la partecipazione dei disabili alla vita sociale ed economica del Paese. Tutto ciò ovviamente ha bisogno, oltre che di attenzioni e di grandi dichiarazioni in merito all'efficienza dell'amministrazione pubblica, anche di finanziamenti.

attraverso questo tipo di tecnologie che nel 2000 ha iniziato a fare politica un italiano, che oggi non c'è più, che si chiamava Luca Coscioni, grazie al quale si è riusciti a far scoprire in questo Paese non soltanto l'esistenza di chi è disabile, ma anche la necessità di far progredire la ricerca scientifica in modo libero. Tutte cose che, se fossimo stati dietro a chi era al Governo o in Parlamento in quegli anni, non avremmo sicuramente potuto guadagnare. Certo, abbiamo guadagnato una reazione di tipo teocratico, che ancora oggi caratterizza le gerarchie vaticane, e anche buona parte delle Aule del nostro Parlamento; ma gli italiani

ma che ha avuto importantissimi riconoscimenti anche dal punto di vista giurisdizionale. La ministra Turco aveva stabilito che tutto questo potesse essere finanziato con 10 milioni di euro. Si tratta quindi di apportare delle modifiche al cosiddetto nomenclatore tariffario e finanziare finalmente la possibilità per decine di migliaia di cittadini italiani di parlare, di avere diritto di parola relativamente a ciò che loro accade come individui psicofisicamente intesi, ma anche come soggetti detentori di diritti.

sarà dare la possibilità agli individui, tanto quanto alle associazioni che rappresentano i disabili, di avere accesso alla RAI-Radiotelevisione italiana, servizio pubblico.

che, mancando l'organo di vigilanza, non è tenuta ad adottare i regolamenti che consentano a tali associazioni, al pari delle tribune politiche organizzate durante l'anno, di avere accesso alla radio

Convenzione internazionale abbiamo scoperto che il Governo ha deciso di tradurre

sottolinea che «ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una responsabilità propria per la promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dai Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali». Si riconosce pertanto questa responsabilità di tutti gli appartenenti

«Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità». afferma che: «Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possano ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri». Ebbene, il nostro Governo

rappresentato in termini di unità all'interno di questo *soviet* supremo della disabilità, ma non gli si dà nemmeno la possibilità di eleggere

dire la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Quest'ultima, all'articolo 20, creava un Fondo nazionale per le politiche sociali.

ma anche economiche e sociali che si frappongono al pieno godimento dei diritti dei disabili in Italia, con la creazione di questo Osservatorio mi

l'ordine del giorno presentato dai colleghi del Partito Democratico e gli emendamenti presentati dalla delegazione radicale dello stesso il Governo dia un segnale di discontinuità.

per depositare gli strumenti di ratifica o comunque per annunciare i tempi certi che sarebbero stati utilizzati per incorporare questa Convenzione nella nostra legislazione. Spero che adesso si faccia tesoro anche delle

si assumano scelte volte ad applicare queste misure internazionali nel nostro sistema nazionale, di segno diverso rispetto a tutto ciò che, invece, ha caratterizzato le politiche sociali e sanitarie di questo Governo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'atto di ratifica che ci apprestiamo a compiere, purtroppo ad oltre due anni di distanza dall'adozione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite e a quasi due anni dalla firma apposta il valore particolare degli atti che sanciscono diritti di uguaglianza e di non discriminazione, e dunque il valore della democrazia. esso deve essere valorizzato per la portata politica e culturale che riveste, vincolando i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione e i Parlamenti che la ratificheranno ad operare per la piena attuazione dei diritti chiaramente affermati delle persone con disabilità, che con disabilità, che nel mondo sono oltre 650 milioni. La Convenzione muove dal superamento del modello medico assistenziale, che considera la disabilità come malattia, e pone al centro la protezione e la promozione sociale del disabile, basata sull'affermazione piena dei diritti umani della persona, vincolando gli Stati ad assumere impegni politici, economici ed organizzativi volti ad assicurare il rispetto della dignità, il diritto all'autodeterminazione e all'affermazione di sé delle persone con disabilità. I contenuti specifici della Convenzione sono già stati richiamati da alcuni colleghi, per cui non intendo ritornarci. Sottolineo piuttosto che in molti Paesi la portata innovativa, quasi rivoluzionaria, dell'affermazione di tali diritti restituisce la cifra della distanza esistente tra la condizione di quei popoli e l'attuazione dei fondamentali diritti di libertà e di uguaglianza. Bastano pochi numeri per restituire questa dimensione: cento dei disabili vive nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo, nei quali, complessivamente, solo il 2 per cento delle persone con disabilità ha accesso all'assistenza, alla riabilitazione, ad un'istruzione formale; sul totale della popolazione disabile mondiale solo meno del 20 per cento accede al lavoro. Nel nostro Paese l'adesione alla Convenzione dovrebbe rappresentare solamente la cornice di un quadro che si è andato componendo nel tempo, a partire dalle grandi riforme sociali e sanitarie degli anni

n. 328 del 2000 hanno tracciato un percorso non solo tra i più completi ed avanzati nell'affermare i diritti delle persone con disabilità, ma hanno definito un approccio culturale, quello della universalità dei diritti, che ci si augura non sia mai messo in discussione. Non ci attendiamo, quindi, dalla ratifica una modifica dell'ordinamento, ma l'impegno alla piena attuazione di quanto il nostro ordinamento prevede. In quest'ambito, infatti, restano molte cose da fare e permangono molte preoccupazioni, non superate dal disegno dal disegno di legge di ratifica in esame. Pochi sguardi sulle condizioni materiali di vita delle persone disabili nel nostro Paese sono sufficienti a mettere in evidenza, ad esempio, i gravi deficit di accessibilità e le gravissime limitazioni alla mobilità che caratterizzano ancora tutto il nostro territorio, i luoghi pubblici - a partire da quello in cui sediamo - e quelli privati, le città ed i territori rurali. Ma il deficit di accessibilità non è declinato solo sul piano fisico: l'accesso al lavoro, diritto costituzionale e strumento primario per l'esercizio del diritto all'autodeterminazione, alla partecipazione, allo sviluppo dell'autonomia, è consentito a meno del 25 per cento delle persone con disabilità, che siano in condizioni di di esercitare un'attività lavorativa. La preoccupazione sull'accesso al lavoro aumenta, come è evidente, in questa fase di grave crisi economica, con i connessi rischi di esclusione ed impoverimento delle persone con disabilità. Molti altri ostacoli si frappongono ancora alla piena attuazione dei diritti di libertà ed autodeterminazione dei disabili: la legge n. 328 del 2000, di riforma dell'assistenza, è ancora inattuata in uno dei suoi aspetti fondanti, vale a dire la definizione delle condizioni concrete di esercizio dei diritti sociali

per l'avvio probabile del percorso di attuazione del federalismo fiscale in un quadro di norme ancora privo di riferimenti certi, di garanzie rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni ed alle risorse necessarie a finanziarli.

Occorre ad ogni costo, con riferimento all'attuazione della legge sull'assistenza, evitare il rischio di una omologazione al ribasso degli standard di offerta e di qualità dei servizi a supporto dell'autonomia e dell'assistenza alle persone disabili, o anche semplicemente che gli standard di riferimento siano definiti in termini medi. Occorre evitare la realizzazione di uno «stato minimo» a fronte del quale la fondamentale opera sussidiaria della società civile organizzata, delle organizzazioni del terzo del *non* *profit* sarebbe pesantemente depotenziata. Nessun soggetto sociale può, infatti, agire in sostituzione se chi rappresenta i cittadini (cioè lo Stato e le istituzioni) non definisce un quadro certo di analisi del bisogno, di programmazione degli interventi e di determinazione delle risorse necessarie a garantire l'esercizio dei diritti. In questa prospettiva desta preoccupazione anche il quadro delineato dal Libro verde del Ministero del *welfare*, che afferma in maniera pienamente condivisibile la centralità dell'approccio alla persona nella sua globalità, la promozione ed il sostegno alla salute ed alla vita attiva, la prevenzione della disabilità e della non autosufficienza, ma poco o nulla dice sugli strumenti di intervento e garanzia della cura e dell'assistenza. Molto spazio in quest'ambito è attribuito infatti alla promozione della sussidiarietà, ma gli spazi di esercizio effettivo della sussidiarietà orizzontale, in carenza di risorse sono, come ho già detto, assai limitati. Il tema delle risorse rimane poi centrale per garantire l'attuazione dei diritti delineati: sotto questo aspetto il disegno di legge di recepimento non fornisce alcuna garanzia, né definisce orientamenti precisi. A fronte di ciò come non richiamare il recente taglio operato dalla legge finanziaria sul Fondo sociale, per 200 milioni di euro, e il mancato ampliamento del finanziamento del Fondo per la non autosufficienza, coerentemente con quanto previsto dal piano di implementazione definito dal Governo Prodi? I rischi di arretramento delle politiche di promozione dei diritti delle persone con disabilità sono aggravati dai seri problemi introdotti nei bilanci dei Comuni, che si fanno in larga parte carico delle funzioni di assistenza alla persona, della mobilità, nonché dei servizi finalizzati a garantire il diritto allo studio, Comuni Comuni i cui bilanci sono gravati dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa. Il diritto alla cura e all'assistenza non è ancora di fatto tale

da assistenti familiari, le cosiddette badanti, per lo più lavoratrici immigrate in larga parte irregolari sia rispetto alla condizione di soggiorno che rispetto alla condizione di lavoro. Al lavoro delle donne immigrate si aggiunge quello delle donne italiane, sulle quali grava ancora la più gran parte del carico di cura, in assenza di un serio piano di investimenti in infrastrutture sociali, cioè in servizi alle persone e alle famiglie, che solo può garantire piena attuazione del principio di pari opportunità a tutte le donne e agli uomini di questo Paese, anche alle persone disabili. Che dire poi dello stato di arretratezza delle politiche e degli interventi per il cosiddetto «dopo di noi», specchio evidente di quanto poggi ancora sulla famiglia, cioè sulla donna, la responsabilità della cura delle persone con gravi disabilità, del rischio potenziale, soprattutto se accompagnato da "revisionismi" culturali, di riaprire un orizzonte concreto all'istituzionalizzazione delle persone non autosufficienti? Come non intravedere poi rischi di arretramento anche sul fronte dell'integrazione scolastica in presenza di possibili quanto nefaste interpretazioni estensive delle neointrodotte «classi di inserimento», o il rischio di progetti di revisione della riforma psichiatrica, che abbiano come obiettivo non la sua piena attuazione ed attualizzazione, ma la messa in discussione del principio di integrazione sociale delle persone con disagio psichico e di territorialità dei servizi? Appaiono allora assolutamente necessari gli impegni proposti al Governo da alcuni colleghi del mio Gruppo, con un ordine del giorno che chiedo fin d'ora di sottoscrivere, a dare tempestiva e puntuale attuazione all'impegno di promuovere, attraverso un apposito piano di azione, le politiche e le misure - anche economiche -necessarie ad assicurare che i diritti e le libertà dei disabili siano effettivamente riconosciuti e tutelati.

Signor Presidente, concordo con quanti mi hanno preceduto ed hanno sottolineato il valore straordinario di questa ratifica, a due anni dalla sottoscrizione

che va sì a vantaggio delle persone con disabilità, ma anche a vantaggio dell'intera società. La conquista dei diritti delle pari opportunità

favorì di fatto una prima e decisiva tappa per affermare il cammino dell'inclusione sociale delle persone con disabilità psicofisiche. Quel movimento ha cambiato la vita di tante bambine e bambini disabili, ai quali per la prima volta fu riconosciuto il diritto di esistere, di essere curati, di essere istruiti,

infatti, la maggior parte di questi bambini e bambine restava chiusa tra le pareti domestiche, nascosta dalle famiglie che si vergognano di loro, privata di ogni istruzione e di ogni cura adeguata ai loro bisogni, oppure veniva chiusa in un istituto dove spesso l'inedia e l'abbandono li portava ad una morte prematura. Da quel momento non solo è nato un rispetto nuovo per i diritti di queste persone, ma la loro diversità, i loro tempi, i loro bisogni diversi, la loro affettività hanno costretto le famiglie, la scuola, la società a crescere e ad arricchirsi socialmente e culturalmente, a cambiare le proprie organizzazioni. La medicina e la scienza sociale e psicologica si sono arricchite di nuovi capitoli.

e questo è avvenuto molto spesso nella disattenzione generale e senza la possibilità di tirare le fila, di fare una verifica condivisa degli obiettivi nel frattempo raggiunti. Oggi, la ratifica da parte del Parlamento italiano di questa Convenzione è quindi una grande occasione per rilanciare un impegno, che è quello di attuare politiche di pari opportunità per le persone disabili e con sottolineo "con" - le persone disabili, nello spirito dei principi proclamati dalle Nazioni Unite, principi che riconoscono la dignità inerente, il valore e i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo. Fatto importante è che in questa Carta si riconosce che la disabilità è un concetto in evoluzione e questa evoluzione c'è stata: l'esempio più eclatante è quello del giovane Pistorius, che corre con le gambe artificiali. Egli ha costretto chi governa lo sport, e non solo chi governa lo sport, ad interrogarsi su quanto quell'ausilio possa essere stato determinante per il raggiungimento di un record sportivo, ma anche a chiedersi in che misura quel risultato sia stato, come è evidente, non solo frutto dei materiali sofisticati con cui è stato costruito l'arto, ma soprattutto il risultato combinato delle tecnologie con le risorse umane, intellettuali e della volontà

Se la disabilità è un concetto in evoluzione, se la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali e ambientali, che impediscono la loro piena ed efficace partecipazione nella società sulla base di parità con gli altri, è chiaro che occorre intervenire su questo, che occorre agire non solo per limitare le minorazioni, ma anche per abbattere le barriere, in particolare quelle ambientali nel senso ampio del termine, che ancora oggi si frappongono al raggiungimento dei diritti e delle pari opportunità. Ciò consentirebbe di favorire l'evoluzione del concetto di disabilità, non perché essa si possa eliminare, ma perché attraverso un'evoluzione positiva si può realizzare una grande crescita per chi è disabile e per la società. Perché questo avvenga non si può solo attuare un atto, per quanto importante, di ratifica. Credo sia significativo il metodo di controllo che viene istituito a livello internazionale per monitorare i risultati raggiunti dagli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione, che mi pare innovativo ed efficace. Occorre che anche a livello nazionale si pongano le basi, come previsto dalla Convenzione, perché i contenuti di questa ratifica si realizzino e si attuino quindi monitoraggi per meglio individuare e valutare i risultati raggiunti e le difficoltà incontrate. Siamo, signor Presidente, in una sede politica istituzionale e credo che le forze politiche dovrebbero prendere atto che è importante anche per la politica e le istituzioni cambiare il modello di progettazione, di elaborazione e di riferimento. Il fatto che ci sia chiesto di includere nelle politiche ordinarie i temi della disabilità è proprio la bussola per determinare questo cambiamento anche nel modello organizzativo e di lavoro delle forze politiche e istituzionali. Si creano in questo momento condizioni importanti e vorrei riferirmi soprattutto ad un punto, prima di concludere, quelloche riguarda il diritto alla salute, che è particolarmente sottolineato all'articolo 25 della Convenzione. Esso è importante in quanto afferma che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Ciò significa porre un obiettivo alto che anche il nostro Paese faticherà a raggiungere, pur avendo un buon Servizio sanitario, in primo luogo perché le diversità nella qualità e nella quantità dei servizi, Regione per Regione, sono ancora troppo pesanti; in secondo perché diversificano così l'esigibilità dei diritti su base regionale; infine perché il nostro sistema è ancora organizzato per dare risposta alla malattia acuta più che alle forme di disabilità, cronicità e agli stadi degenerativi. Se la salute è prevista come un diritto e se la salute è considerata il benessere complessivo della persona e non solo l'assenza di malattia, mi duole sottolineare - ma purtroppo così è - che i tagli fatti al Fondo sociale, a quello delle politiche familiari e dal 2010 anche sui fondi della sanità renderanno più difficile il raggiungimento di questi obiettivi. Il valore universale di queste conquiste, che mettono in piena luce le discriminazioni che oggi colpiscono soprattutto i bambini e le donne disabili, più soggetti di altri a violenze e vessazioni,

- su questo credo che sia importante la nostra attenzione - di coinvolgere tutti quei soggetti che nel Paese operano su queste tematiche, anche le forze politiche e sociali. Il punto è che l'osservatorio svolga la sua azione in un contesto che affermi il criterio della sussidiarietà, ma anche che informi annualmente il Parlamento del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti. Solo così

di parità effettiva e concreta affinché queste persone possano partecipare alla pari di tutti gli altri alla vita sociale del nostro e degli altri Paesi. Una Convenzione che rispecchia nei principali temi - l'istruzione, il lavoro, l'inclusione sociale, la politica culturale ed economica, finanche lo sport e lo svago - la legislazione italiana e su tale impostazione hanno convenuto convenuto tutti i 192 Paesi aderenti alle Nazioni Unite. L'Italia, purtroppo, a causa dell'anticipata fine della scorsa legislatura non aveva ancora provveduto alla ratifica della Convenzione. Una Convenzione che costituisce un importante obiettivo raggiunto dalla Comunità internazionale, in quanto fino ad oggi non esisteva in materia di disabilità uno strumento internazionale vincolante per gli Stati, se si escludono appunto le Regole standard dell'organizzazione delle Nazioni Unite sulla disabilità, che risalgono al 1993 e che comunque sono prive di efficacia vincolante. Perché è importante? Il raggiungimento di tale obiettivo dà concretezza a quella che era un'utopia delle persone con disabilità: essere, esistere, vivere alla pari delle opportunità di tutti. E la Convenzione, infatti, non introduce nuovi diritti, piuttosto si prefigge lo scopo di promuovere, proteggere ed assicurare alle persone con disabilità il il pieno e uguale godimento del diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, ad una vita indipendente, alla mobilità, alla libertà di espressione e, in generale, alla partecipazione attiva alla vita politica e sociale. Sono gli obiettivi che vedono impegnata fin dalla sua costituzione l'Associazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca scientifica, che con il suo fondatore, Luca Coscioni, da politico e con un corpo malato di sclerosi laterale amiotrofica, ha posto l'urgenza della liberazione del malato o del disabile da ogni forma di discriminazione, emarginazione, esclusione o restrizione dei diritti umani civili e politici.

Severino Mingroni ha inviato al Presidente del Consiglio dei ministri un video per mostrare come vota un disabile,

Le critiche le abbiamo fatte e le rifaremo comunque, perché, pur credendo nell'importanza e avendo lottato da anni perché questa Convenzione dell'ONU venisse ratificata, ciò nonostante è anche giusto parlare di quei punti

che appare più simile alle solite sovrastrutture che si sperava di non vedere più piuttosto che ad un organismo efficace e competente. Però, di questo riparleremo anche in occasione del voto degli emendamenti proposti dalla delegazione radicale nel

il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità».

che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica

che vuole occuparsi di corpi da mantenere obbligatoriamente in uno stato di non vita grazie alle macchine, non vuole che quelle stesse macchine, quella tecnologia, quella scienza, quella ricerca siano

disabilità. Altrettanto curiosamente, in occasione della Giornata della memoria, il Vaticano, il Papa, con una coincidenza che ha dell'incredibile, ha riabilitato i lefebvriani, cioè coloro che negano l'Olocausto.

ratifica la Convenzione sulla disabilità. Io credo che dovremmo domandarci quando dedicheremo una seduta al dibattito sui rapporti che manteniamo con questo Stato

Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Sottosegretario, oggi per noi è una giornata molto importante: accettiamo un impegno determinante: quello di abbattere tutte le barriere architettoniche, sia fisiche sia culturali, verso le persone diversamente abili.

Certamente le pressioni del mondo internazionale hanno portato - direi finalmente - a porre al centro dell'agenda politica la ratifica della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone disabili. Ricordiamo che tra i primi a firmare questa Convenzione siamo stati noi, il Governo Prodi nel 2006,

Si stima che nel nostro Paese vivano circa 3 milioni di persone disabili, cioè il 4,8 per cento della popolazione. Siamo di fronte a statistiche riportate nel 2005 dall'ISTAT. A dare un quadro più recente, del 2007, ma anche più forte e completo, è l'Eurostat, Ufficio di statistiche dell'Unione europea, il quale ha calcolato che sulla popolazione europea tra i 16 e 64 anni le persone disabili in Italia sono il 6,6 per cento e più precisamente oltre 4 milioni. Non va dimenticato che stiamo parlando di una fascia in età

il compito di far entrare l'Italia nella comunità internazionale che tutela tutti i diritti dei disabili con i fatti e che cerca di migliorare le condizioni di 650 milioni di persone disabili in tutto il mondo, proprio perché non è un atto banale e perché è un atto che vincola tutti gli Stati che lo sottoscrivono. La Convenzione, come stabilisce l'articolo 1, vuole promuovere, proteggere e assicurare alle persone con disabilità il pieno ed uguale godimento del diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, a una vita indipendente, alla mobilità, alla libertà di espressione e, in generale, alla partecipazione attiva alla vita politica e sociale. Come è evidente, non si stabiliscono nuovi diritti, ma scopo della Convenzione è garantire la piena affermazione di tutti quei diritti che sono scritti nelle Costituzioni, e in quella italiana in modo ancora più efficace, ma che spesso purtroppo non trovano la giusta forza per essere affermati. Per questo, siamo di fronte ad un documento che si occupa esclusivamente e totalmente di disabilità e vincola a dare maggiore forza e maggiore applicazione al sistema dei diritti dei disabili con tutte le peculiarità che ne concernono, considerando che si vuole consolidare che le persone con disabilità godano degli stessi diritti degli altri cittadini, che abbiano finalmente delle pari opportunità. In tutti gli articoli della Convenzione ONU si punta su questo principio e non è un caso che proprio l'articolo 1, al comma 2, sancisce un concetto cardine: l'abbattimento delle barriere, di tutte quelle barriere non solo fisiche ma anche culturali, mettendo in luce che la disabilità esiste perché esistono le barriere, che sono ostacoli che sono ostacoli per tutti i portatori di minoranze fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali di lunga durata, i quali hanno comunque il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla vita della società.

una delle azioni quotidiane, come mangiare o vestirsi. È fondamentale tener presente che deambulare è un diritto umano: questo è un principio che la Convenzione dell'ONU afferma con estrema chiarezza. Ora, la ratifica della Convenzione impegna le 192 Nazioni che compongono l'Assemblea generale dell'ONU ad adottare leggi che proibiscano discriminazioni basate su qualsiasi forma di disabilità, eliminando dalle loro legislazioni ogni norma o provvedimento discriminatorio verso le persone disabili. Il nostro, il mio auspicio è che oggi una delle nostre vere priorità sia combattere luoghi comuni e pregiudizi, valorizzando il ruolo e il contributo dei cittadini con disabilità. Una particolare attenzione è richiesta nei confronti di donne e bambini, che hanno certamente una maggiore difficoltà e vulnerabilità. Verso le donne con disabilità viene riconosciuto, con l'articolo 6, l'impegno affinché ogni Stato adotti ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo, l'avanzamento e il rafforzamento della loro condizione. Allo stesso modo, una protezione maggiore deve essere rivolta verso i bambini, che devono essere tutelati e protetti, sia all'interno della famiglia, sia all'interno della scuola e della società. A loro gli Stati devono garantire (secondo quanto è richiamato all'articolo 7) il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri bambini. non vengono sottovalutate l'istruzione, la formazione professionale e la salute. Con la ratifica di questa Convenzione, tutte le scuole e i luoghi di educazione dovranno prevedere l'integrazione scolastica, con il supporto individualizzato, in grado di incidere sul progresso scolastico e, soprattutto, sulla socializzazione garantendo loro così (in base a quanto stabilito dall'articolo 24) la formazione professionale e l'ingresso ai sistemi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita; senza lasciarle sole nel periodo lavorativo, perché compito degli Stati è riconoscere il diritto delle persone con disabilità, su basi di parità con gli altri, anche attraverso la costruzione di un mercato del lavoro

La Convenzione si radica inoltre nella convinzione che la discriminazione delle persone sulla base della disabilità sia una violazione della dignità della persona umana e nella consapevolezza che, nonostante i vari strumenti legislativi, le persone con disabilità continuano ad affrontare ostacoli nella loro partecipazione come membri della società e violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo. Non si può, a questo punto, essere il lavoro che la 3ª Commissione ha portato avanti in maniera veloce e snella, con il doveroso e prezioso contributo dell'opposizione, testimonia come siamo di fronte ad obblighi universali e condivisi, oltre che internazionali. Su tre aspetti, comunque, vorrei concentrare l'attenzione di noi senatori. il principio dell'accessibilità, che viene richiamato nella Convenzione all'articolo 9, il quale sancisce il principio secondo cui le persone con disabilità hanno il diritto di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita. In base tutti gli Stati sono tenuti ad adottare tutte le necessarie misure per assicurare l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione, alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Questo deve farci chiedere anche quanto tutto ciò sia oggi possibile nel nostro Paese. "Fruibilità" e "accessibilità" devono diventare termini propri del linguaggio di ogni opera pubblica e privata che si vuole realizzare. A parte la praticità, è importante raccogliere anche l'esigenza di un disabile, che non è solo quella di vestirsi, mangiare o uscire. Non ci sono soltanto le esigenze primarie, ma c'è anche quella, per esempio, di divertirsi, di visitare un museo, di poter andare al parco, allo stadio, al teatro o al cinema come uomo e non come disabile. Anche la fruibilità è il superamento dell'indifferenza, perché vuol dire "usabilità", cioè la possibilità effettiva di utilizzazione agevole e sicura dell'ambiente in favore dell'uomo, un ambiente che comprende tutti gli spazi racchiusi e naturali e l'utilizzazione delle relative attrezzature e dei servizi offerti. Un altro punto su cui vorrei venisse focalizzata l'attenzione è la costituzione dell'Osservatorio nazionale

con uno stampo burocratico, in cui le associazioni dei disabili alla fine non trovano vera rappresentanza.

sia veramente incredibile che i fondi su cui grava l'Osservatorio in questione siano quelli per i servizi sociali. È per questo che non vorrei che la ratifica di questa Convenzione restasse solo un atto isolato, un impegno internazionale a cui il Governo non fa seguire i giusti interventi finanziari. In tal senso, vorrei raccogliere

per la finanza pubblica, le esigenze di sostegno e di supporto delle persone con disabilità e dei loro familiari non devono essere sottovalute.

infine ricordare tutti coloro che, professionisti e volontari, lavorano nei servizi pubblici, nelle associazioni, nelle organizzazioni sociali e nelle fondazioni, occupandosi delle persone diversamente abili. Mi piace concludere il mio intervento ricordando le parole di Oscar Pistorius che, in prossimità delle scorse Olimpiadi, ha detto: «Vorrei correre in pista e nella vita come uomo e non come uomo senza gambe».

ringrazio innanzitutto il sottosegretario Mantica per la sua presenza. «Niente su di noi senza di noi»: è molto più di uno slogan del movimento globale delle persone con disabilità; è la consapevolezza della disabilità quale partecipazione attiva alla società; è una denuncia contro le barriere materiali, psicologiche ed architettoniche che ancora coinvolgono i portatori di handicap senza possibilità di ascolto. Prima di cambiare i nostri edifici, di rendere agibili le strade, di permettere gesti che per le persone che non hanno handicap appaiono banali - e questi gesti sono sicuramente molto importanti - occorre però cambiare la mentalità, togliere il pregiudizio e riuscire a guardare tutto ciò che ci circonda con occhi diversi, gli stessi di chi si affanna nel salire un gradino o prendere un mezzo pubblico. La Convenzione delle Nazioni Unite e il Protocollo attuativo sui diritti delle persone con disabilità sono un passo importante, oserei definirli un atto di civiltà che è entrato in vigore, in quanto ratificato da 20 Paesi sottoscrittori, il 3 maggio 2008. È il primo grande Trattato sui diritti umani del XXI secolo, colmando una lacuna nel diritto internazionale. La Convenzione, con i suoi 50 articoli, elabora in dettaglio i diritti delle persone con disabilità, occupandosi di diritti civili e politici, accessibilità, partecipazione, diritto all'educazione, alla salute, al lavoro e alla protezione sociale; soprattutto, la Convenzione riconosce che un cambiamento di atteggiamento nella società è indispensabile per consentire alle persone con disabilità di raggiungere la piena eguaglianza. Sebbene, infatti, soprattutto in Paesi come l'Italia, la Costituzione garantisca in principio gli stessi diritti per tutti, in pratica sappiamo - lo sappiamo noi che facciamo politica, ma lo sanno soprattutto le famiglie che hanno al loro interno persone che vivono una condizione di disabilità - che i disabili incontrano discriminazioni in tutti gli aspetti della vita quotidiana (il lavoro, l'educazione, la salute, l'esercizio dei loro diritti), eppure contribuiscono alla società in un'infinità di modi e contribuirebbero ancora di più se fossero pienamente integrati nella comunità. La dignità di circa il 10 per cento della popolazione mondiale, pari a 650 milioni di persone affette da disabilità, non può essere ignorata, ma è un diritto che va ribadito e concretizzato nella vita civile, culturale, economica, politica e sociale. Il testo base di ratifica sottoposto al nostro esame prevede uno strumento in più rispetto ai 50 articoli della Convenzione, cerca di coniugare anche i princìpi contenuti nella legge n. 104 del 1992, cui facevano riferimento alcune colleghe che sono intervenute, e introduce l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che ha il compito di promuovere la piena integrazione delle persone disabili

Tuttavia, c'è un aspetto che vorrei porre all'attenzione dell'Aula riguardante, in particolare, la salute riproduttiva. Gli articoli 23 e 25 contemplano il giusto e positivo obiettivo della persona disabile di far famiglia e di poter godere di tutte le cure sanitarie. Esprimo invece una perplessità sul fatto che la disabilità del feto possa essere ritenuta una precondizione per offrire e ricorrere all'aborto. La ricerca della perfezione, lo dico umilmente, credo sia un po' un'ossessione della nostra società mal si identifica con il valore della vita umana che contiene nel suo valore intrinseco e antropologico l'essere stesso della non perfezione assoluta. In fondo, si rischia quasi di travolgere il diritto a vivere, che raccoglie l'essere umano nella sua ricchezza e nelle sue debolezze e imperfezioni. Non possiamo credere in una sorta di selezione naturale dove il debole, il fragile, l'imperfetto, così come ai tempi di Sparta, non è degno di venire al mondo, attuando di fatto una selezione eugenetica. Questa Convenzione esprime la giusta e corretta volontà di proteggere le persone con disabilità; è quindi difficile coniugare l'importanza del disabile nella società, la tutela della diversità e poi sancire una sorta di blocco al momento della nascita. Positivo, però, è che per la prima volta la Convenzione riconosca una specificità di genere

I verbi elaborati in questo lavoro preparatorio sono: promuovere, proteggere, garantire, riconoscere, includere, rispettare, valorizzare. Io li definisco i verbi della speranza per le persone diversamente abili, ma anche per quelle abili, perché una comunità veramente civile non può e non deve operare nessuna forma di discriminazione manifesta o subdola. Ogni persona è unica e irripetibile, porta in sé quella ricchezza che contribuisce a realizzare un mondo migliore. L'importanza della Convenzione attraverso la ratifica che oggi approviamo insieme al Protocollo rappresenta un importante passo in avanti non di un singolo Stato, ma dell'intera comunità mondiale. I 20 Stati che per primi hanno ratificato la Convenzione

i principi sono affermati con chiarezza, però troppo poco la politica si spende per rendere esigibili i diritti. L'obiettivo, quindi, è quello di far crescere una cultura del rispetto, oserei dire dell'amore, della fraternità, capace di accogliere tutti, per superare le discriminazioni e realizzare politiche di uguaglianza. Credo che questa Convenzione sia la traduzione politica di un principio universale, la regola d'oro: «Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te». Con questo brocardo si pongono in essere i tre valori fondanti lo Stato moderno, quali la libertà, l'uguaglianza e la fraternità. Ma soprattutto attraverso l'attuazione di un principio elementare nella forma, ma non nel contenuto, l'uguaglianza di aspettative si tradurrebbe in uguaglianza di diritti. Concludo dicendo: diversi ma uguali.

mi atterrò all'illustrazione dell'ordine del giorno che assieme ad altri colleghi ho presentato per accompagnare l'approvazione di questo provvedimento. Un ordine del giorno che, innanzitutto, riepiloga le ragioni per cui arriviamo con un certo ritardo ad adempiere ad una promessa fatta alle associazioni delle persone disabili e che - ricordo - congiuntamente al Governo hanno firmato nella sede delle Nazioni Unite assieme a noi

le associazioni dei disabili sono state protagoniste in prima persona della ridefinizione dei loro diritti e delle loro tutele in campo mondiale e internazionale. Arrivare oggi, con un certo ritardo, alla ratifica

che all'inizio di questa legislatura il Governo abbia ridotto, fino a cancellarli, gli stanziamenti a favore del fondo per le persone non autosufficienti.

dei gradi di disabilità, facendo leva soprattutto sulla residua capacità di vita autonoma, che è il principio ispiratore della Convenzione: si deve cioè consentire ad ognuno di rimuovere quegli ostacoli che gli impediscono non solo di avere pari opportunità, ma di vivere pienamente una vita autonoma e dunque di non dipendere in maniera prevalente da chi gli sta intorno o da interventi di natura assistenziale.

bisogna stare molto attenti, perché queste discriminazioni sono sempre dietro l'angolo, magari perché ci si spiega che si vuole attuare sistemi più semplici, più governabili di una condizione che invece mette tutti noi di fronte a situazioni di difficoltà alle quali bisognerebbe rispondere non solo con la testa ma anche con il cuore, con intelligenza e con la capacità di fare società e solidarietà. Poi, vorremmo - e questo è il senso del nostro ordine del giorno - accompagnare questa Convenzione con la predisposizione di un Piano d'azione che abbia tempi e priorità cadenzate e che sia sotto la responsabilità del Governo, non di un Osservatorio che non ha né tempi né vincoli per presentarlo. Quindi, un atto impegnativo del Governo, portato all'attenzione del Parlamento, e un atto del Governo che consenta anche di verificare nella sua concretezza

molto perplessi sulla ridondanza di questo strumento, e la prevalenza al suo interno dei rappresentanti ministeriali su quelli delle associazioni e delle famiglie delle persone disabili scompensa disabili scompensa la capacità di costruire un volano vero di attuazione di politiche e di priorità, dando più una soluzione burocratica al problema, che non di tempestività e di azione concreta. Quindi, con l'ordine del giorno G100 si chiede al Governo di mettere accanto alla ratifica della Convenzione, di questo atto così importante, gli strumenti e la partecipazione del Parlamento al monitoraggio della sua attuazione,

Per questa ragione è utile che il Parlamento abbia la possibilità di continuare a seguire, su predisposizione di atti e pareri di Governo, la concreta attuazione di questa Convenzione

Signora Presidente, intervengo su un aspetto specifico del disegno di legge di ratifica, in particolare su un aspetto che il Governo

e per il modo in cui il Governo, complessivamente, recepisce la materia. Nel momento in cui si opera una deviazione rispetto alle procedure giuridiche normali,

calcare la mano sulle effettive difficoltà che la persona disabile può manifestare; si sottolineano, invece, le potenzialità che la persona disabile

anche perché - mi rivolgo al rappresentante del Governo sperando abbia la bontà di ascoltare - dagli anni Novanta è stato istituito presso il Ministero dell'istruzione un Osservatorio nazionale sull'handicap che ha lavorato per molti anni con le università

e senza portare avanti alcun intervento massiccio di formazione qualitativa. Credo dunque sia assolutamente necessario che il Governo dia, almeno in questa sede, visto che non ha prodotto alcun emendamento nella fattispecie, un segnale di apertura,

non è detto che una persona paraplegica non possa prendere una laurea in qualunque disciplina; non è detto che una persona che oggi ha alcuni problemi in futuro non possa risolverli e quindi arrivare alle più alte sfere dell'istruzione e della formazione. È scritto nella nostra Costituzione repubblicana che lo Stato rimuove gli ostacoli che si frappongono a tutto questo. Credo che mai parole siano state più sagge e che mai come adesso esse debbano essere recepite da un Governo che vuole e deve dimostrarsi sensibile

rispetto alle diverse disabilità, che vanno considerate nella loro tipicità, o per meglio dire atipicità, perché sarebbe un capitolo a parte, su cui probabilmente dovremmo anche svolgere una riflessione come opposizione, ma soprattutto come maggioranza, nel momento in cui si va a toccare la scuola così come è stata toccata. Piuttosto, chiederei al Governo di esprimersi se almeno c'è la volontà di recepire quanto noi come Partito Democratico stiamo proponendo, perché credo che questa sia una lacuna vistosa e pesante,

Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, nel maggio del 2008 è entrata in vigore la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. È un faro, che illumina le politiche nazionali in materia di disabilità. In Italia sono calcolati circa 3 milioni di disabili, come ha riferito la collega poc'anzi, il cui numero, considerando anche gli affetti da problematiche più lievi, certamente si raddoppia. Nel mondo ne sono stimati circa 650 milioni. La Convenzione che ci apprestiamo a ratificare nasce dalla necessità di dare attuazione vincolante per gli Stati contraenti alla tutela dei diritti di pari opportunità e non discriminazione dei disabili. L'allarmante constatazione della negazione dei diritti umani genera il forte richiamo dell'ONU affinché le politiche determinino una reale integrazione. I percorsi culturali della nostra formazione ci hanno portato, a seconda delle stagioni della vita, a guardare talvolta con ammirazione le leggi di Sparta e tal'altra a sentirci feriti, come ieri, nella commemorazione della Shoah, per le follie senza limiti che hanno determinato nel non lontano 1939 l'«operazione T4», per la soppressione dei disabili, degli imperfetti, dei malati, degli esseri improduttivi. Dall'orrore del rifiuto sociale violento corre veloce la nostra attenzione alle generosità che il secolo scorso medesimo è stato capace di offrire: le attenzioni e le braccia aperte di Don Gnocchi, la capacità di formare e accogliere di Don Orione e - perché no? - la disponibilità all'accoglienza illimitata del Cottolengo. Sono i casi estremi dell'odio e dell'amore che scandiscono la storia di eventi straordinari, perché la società ha provato, e forse ancora prova difficoltà a ritenere storia ordinaria la vita di un disabile. Nel preambolo della Convenzione vi è un intero alfabeto di note che stigmatizzano discriminazioni, violenze, permanenza di ghetti culturali ancora legati a «razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione». In uno stadio ideale della vita dobbiamo far sì che nelle sfide quotidiane tutti abbiano la possibilità di vincere, di sognare e raggiungere un traguardo. Le politiche di inclusione e di condivisione devono fare in modo che l'incontro con la disabilità, con la sofferenza divenga un arricchimento capace di coinvolgerci in un futuro comune, dove si possegga un diritto già acquisito: la serenità, la non violenza, senza carità pelose, ma proprie di un costume e di una cultura della reciproca promozione. Spesso lo Stato distratto ha rivolto lo sguardo altrove e per fortuna il volontariato ha coperto ampi settori di silenzio della società organizzata, per andare incontro con interventi prima sul singolo e poi sulla famiglia. Vi è stata una gara indubbiamente di generosità, ma sicuramente inadeguata rispetto alle reali esigenze di una politica guidata da una logica assistenzialistica. Gli stessi disabili sono stati plasmati da questa scuola e spesso è sembrato che ci chiedessero solo questo. È ancora alta l'esclusione sociale legata alla disabilità, il disabile ancora non può essere se stesso, per un "io" che percepisce umiliazioni, difficoltà, barriere. Esclusione e discriminazione sono l'esito di pregiudizi, di cecità culturale. La Convenzione in oggetto ha l'ansia indubbia di eliminare la diversità dal vocabolario delle nostre percezioni e vuole essere lo strumento affinché mai più, culturalmente, essa sia inferiorità. Abbiamo incontrato nella storia esempi simbolo di successo oltre l'infermità e forse per un attimo abbiamo pensato che potesse divenire un messaggio di superamento della emarginazione per la possibile e dovuta integrazione: ieri Roosevelt con la sua poliomielite, con la sua sedia a rotelle è riuscito a guidare una grande Nazione, ad avere un ruolo mondiale. Oggi Pistorius, tanto citato in questa mattinata. Il «*Time*» lo riporta tra i 100 uomini più influenti del pianeta, tra i personaggi il cui potere, il cui talento o il cui esempio morale sta trasformando il mondo. È la voce data dai *media* ai bisogni silenti, agli anonimi problemi di quotidianità drammatica. Nella mia vita professionale tra questi due estremi simboli positivi ho incontrato nelle sale operatorie il cingalese poliomielitico o spastico da mettere in piedi e il poliomielitico delle ultime infezioni delle campagne meridionali che hanno avuto attraverso la medicina ed il percorso del volontariato la possibilità di non essere esclusi e sia pure parzialmente recuperati abbandonando un letto o una sedia. Oggi tecnologia e medicina con informatica e biotecnologia realizzano ausili e protesi che interagiscono con il corpo e con la mente. Vi sono creazioni che hanno già reso antico il *facemouse* o l'*eye tracking* con macchine che utilizzano la forza del pensiero. È sufficiente questa risposta scientifico-tecnologica della società? Ma a quanti assicuriamo la possibilità di conoscere e accedere a questi dispositivi per l'inserimento sociale? Per quanti legiferiamo onde favorire l'incontro con la tecnologia e poter realizzare l'orizzonte primario della persona, la soggettività? Gridiamolo in questa Aula per noi ma anche per tutti quei 650 milioni che non possono farlo. La Convenzione che ratifichiamo e l'Osservatorio che approviamo servono a togliere il dolore di un corpo "pesante" che trova difficoltà a realizzare i propri progetti. Gli ausili modificano la vita del soggetto disabile ed anche di chi gli è intorno. Ne trasformano le relazioni. La casa ha già per i fortunati tecnologizzati una dimensione e funzionalità diversa ma deve averla anche nella organizzazione psico-sociale per non determinare nuovi abbandoni. La Convenzione impegna gli Stati anche con l'accesso alle tecnologie a garantire una vita indipendente, libera, sicura, con pieni diritti di cittadinanza e di tutela della salute, cercando il diritto non al minimo ma al massimo delle possibilità sociali. Nell'attenzione e nella trasformazione sociale, la cultura riabilitativa italiana ha avuto il merito di produrre grandi sforzi per la piena integrazione del disabile. Scuole importanti con nomi che conoscete, come Silvano Boccardi, Cecilia Morosini, Vittorio Valerio, ne hanno prepotentemente valorizzato potenzialità. Da una riabilitazione dedicata al mutilato di guerra, adulto o bambino, ad una vera scuola di inclusione sociale e di recupero alla vita. Spesso il ritorno al lavoro, il ritorno alla capacità di relazionarsi sono sembrati miracoli, ma la forza delle leggi deve far sì che tutto ciò divenga partecipazione ordinaria alla società, alla vita di una famiglia, al recupero pieno di una vita. Sono affetti, relazioni di libertà che devono essere assistite e sono la risposta al «dopo di noi», all'angoscia della preoccupazione dei genitori per il futuro nel quale mancheranno. il Parlamento che ratifica questa Convenzione deve sentirsi coinvolto ad attuare nelle istituzioni ogni politica che garantisca il «dopo di noi». I traumi della strada e del lavoro, gli esiti delle malattie, ciò che improvvisamente rende la vita mai più come prima siano il nostro problema, non solo di chi ha la sorte di incapparvi. I verdetti inappellabili della vita è necessario che siano presi sulle spalle da tutti noi affinché la disabilità che ne è l'esito non sia rifiutata da colui che ne è colpito. Accettiamola noi. La scelta di continuare a vivere è sempre una conquista e lo deve essere oggi per questo Parlamento come per chi si incontra con il disagio improvviso. Scegliamo di essere, non solo in un momento, con gli emarginati, con coloro che non diventeranno mai belli o campioni e trasformiamo le disposizioni di legge in possibilità concrete. Il diritto alla salute ed al lavoro non siano percorsi ad ostacoli. Le attenzioni che hanno determinato l'approvazione di leggi per facilitare categorie cosiddette protette siano momento di attuazione reale, nei pubblici istituti innanzi tutto, e poi anche nelle attività private. Non è una cerimonia o una liturgia quella di oggi, ma è un'emozione coinvolgente l'impegno di ogni parlamentare in questa Aula che ci spinge a confrontarci con le sfide, i dubbi e le prospettive dell'integrazione sui temi della quotidianità. È un modello in cui la nostra comunità si riconosce nelle radici profonde della generosità e della sensibilità che la Convenzione presuppone come forze motrici di un impegno non mediatico ma di amore e di rispetto per la nostra comunità. Nell'agenda politica di questo Parlamento, e conseguenzialmente di questo Governo, c'è il superamento delle barriere e delle frontiere che generano solitudine e angosce ed il recupero dei valori di condivisione sociale delle problematiche dei singoli e delle famiglie, per una politica di inclusione e integrazione. Forse rimuoveremo ai disabili solo molti piccoli ostacoli

il relatore ha ascoltato con molta attenzione gli argomenti che si sono sovrapposti in questa discussione generale

Mi dispiace per i colleghi che hanno attribuito ad una prudenza, se non a una viltà del relatore, l'aver lasciato più spazio alla discussione generale che non alla relazione. Ma i colleghi che erano presenti in Commissione dovrebbero ricordare come il testo originario, del quale fui relatore, era quello, a prima firma della collega Finocchiaro, le firme di tutti i colleghi del centrosinistra, e che un onesto relatore del centrodestra non ebbe alcuna difficoltà a svolgere una relazione che implicava valutazioni favorevoli. Perché le mie valutazioni sono favorevoli? È stato richiamato in molti interventi, da ultimo nelle belle e suggestive espressioni del collega Saccomanno, ma voglio ricordare anche la senatrice Poretti, che questa Convenzione non riconosce nuovi diritti (e non voglio aprire una discussione filosofica se esistano nuovi diritti da dichiarare o vecchi diritti da preservare, perché significherebbe ritornare al 1688 inglese ed al 1789 francese). Quel che è certo, come molti hanno rilevato (con molta precisione anche la senatrice Bianchi), che questa Convenzione, nei suoi princìpi ispiratori, non è fatta per riconoscere diritti alle persone con disabilità, per dischiudere a loro prospettive di crescita nelle politiche di settore, che restano nazionali. Essa si inserisce

come esseri umani, e non come disabili. È chiaro che ciò implica sul terreno degli ordinamenti nazionali politiche di settore, però non si possono sovrapporre i due argomenti. Una delle ragioni per le quali non ho voluto integrare

con la novità ordinamentale dell'Osservatorio, sul quale si sono concentrate le proposte di ordini del giorno e di emendamenti, mi è sembrato che in sede di rapporto tra Parlamento e Governo in occasione delle ratifiche le politiche di settore dovessero restare un passo indietro. Allora, da questo punto di vista - sono sicuro che giustamente colleghi come la senatrice Poretti e il senatore Perduca continueranno a tacciare di eccesso di prudenza il relatore

aveva già fatto, con molta lucidità, la senatrice Bugnano): esso nasce nell'ambito internazionale dell'arco di opinione pubblica dell'associazionismo del mondo dei disabili. L'Italia aveva allora il Governo Prodi e, come lei ha detto risalendo in *flashback* a quando c'era un precedente Governo Berlusconi ed il ministro di settore era, mi sembra, Maroni, il ministro Ferrero - firmatario mi sembra nel marzo 2007 di questa Convenzione, in quanto tra pacchettamenti, spacchettamenti e ping pong non era al vertice di una amministrazione anche ci avesse pensato (mi sembra che, con qualche eleganza, la collega Donaggio abbia alluso al fatto che ci aveva pensato) non avrebbe potuto istituire un organismo del genere di quello introdotto ora dal Governo.

una cura dimagrante rispetto alla ridondanza dell'organismo, mentre noi, senatrice Donaggio, abbiamo entrambi una certa esperienza del rapporto tra gli ordini del giorno e la pubblica amministrazione

del Ministero degli esteri o comunque della pubblica amministrazione, debbono essere individuati nell'ambito dell'associazionismo dei disabili. io dico certamente di sì sul piano delle politiche di settore, così come molte considerazioni che sono state fatte in quest'Aula hanno un senso nell'ambito delle politiche di settore, ma non nel contesto della ratifica di accordi internazionali. In sede di ratifica di un accordo

nel giorno successivo a quello del ricordo della Shoah, e quelle del senatore Saccomanno), non possiamo sovrapporre questi due compiti istituzionali. Sono queste le ragioni per le quali, nell'assoluto rispetto di quella che sarà l'opinione del Governo,

estranei alla valutazione del Parlamento in sede di ratifica. Allo stesso modo, senatrice Poretti, aver richiamato quell'articolo di questa Convenzione come una forzatura di un Ministro che lo ha citato in un atto di indirizzo e coordinamento non mi sembra osservazione pertinente in questa sede. Anch'io mi sono astenuto sia in Commissione sia in Aula dal caricare di profili specifici, sui quali tutte le sensibilità

tradizione liberale e radicale sono portare i diritti umani nel terreno del diritto comune, non del diritto corporato, del diritto speciale o della politica di settore. Ciò non nega valore, attualità, e in alcuni casi intelligenza, agli argomenti che hanno sostenuto la senatrice Sbarbati sul fronte delle politiche della pubblica istruzione o la senatrice Baio sugli aspetti sanitari. concedetemi che ciò che è pregiudiziale dal punto di vista della sanità è che il disabile non può essere usato per la ricerca e questo è quel terreno comune per il quale, nonostante le sue polemiche nei miei confronti, spero di non mancare di rispetto alla tradizione politica che il collega Perduca rappresenta

dire tuttavia, in questo caso sottolineando una inopportunità del Governo, che le ratifiche non dovrebbero mai prevedere l'inserimento di articoli specifici - l'ha già detto molto bene il relatore altrimenti la ratifica diventa un dibattito sul merito dell'accordo, cosa che non dovrebbe essere. Dico questo perché tutto il dibattito in realtà si è svolto intorno all'articolo 3

che poi non è stato approvato per la fine anticipata della legislatura. Voglio ricordare altresì a tutti gli intervenuti che questo Osservatorio non è il frutto o un'invenzione di un atto di burocrazia, ma è il prodotto di una lunga concertazione avvenuta tra l'amministrazione dello Stato e la società civile. l'idea del Governo, che ovviamente a questo punto diventa apprezzabile, di cogliere l'occasione di questa ratifica per inserire l'articolo 3 con l'istituzione di un Osservatorio, su cui già da molto tempo

mesi l'Osservatorio che qui stiamo istituendo sarà il più funzionale e rispondente alle esigenze che sono state avanzate, vi è l'occasione di aprire un'eventuale discussione. Voglio ricordare che spesso il tempo ha un suo valore, anche negli atti parlamentari.

Inserire l'articolo 3 è comunque un impegno ad avere nell'Osservatorio uno strumento e un tavolo di dialogo, di osservazione e di monitoraggio per quanto concerne l'attuazione della Convenzione. Il Governo accoglie quindi l'ordine del giorno,

con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità finestra"), *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo nel presupposto che la che la copertura a valere sul Fondo per le politiche sociali si intenda riferita agli importi in tabella C determinati con la legge finanziaria per l'anno 2009. Esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti».

vorrei aggiungere la firma della senatrice Poretti e la mia all'ordine del giorno G100, che non va nella direzione opposta agli emendamenti testé rigettati dal Senato.

all'occupazione del differentemente abile.

sottolineare come, laddove il disabile sia stato inserito, questi sia stato spesso di esempio per le sue residue capacità lavorative, espresse sempre al massimo delle sue possibilità e come in questo settore la tecnologia ormai risolva o limiti quasi tutte le barriere, infatti non esistono quasi più barriere strutturali, se vi è la Il rischio, signor rappresentante del Governo, è che, in questo periodo di crisi, nei tagli venga anche inserita questa categoria di persone che più di altre ha bisogno di un sostegno.

Così vorremmo misure legislative che prevedano una facilitazione del lavoro del volontariato e del terzo settore, che hanno svolto in questa particolare tematica un ruolo insostituibile. Infine, il Fondo nazionale per le politiche sociali richiamato in questa Aula

Lo avevamo richiesto, senatrice Donaggio, anche al ministro Ferraro, come assessori alla sanità, ma non era stato ottenuto. Così lo chiediamo con maggiore forza a questo Governo:

E, a parte qualche sbavatura forse dipendente dal fatto che i tempi hanno consentito di ampliare la materia, sembrava che su questo tema non si potesse non essere tutti unanimemente d'accordo.

convergessero nel riconoscimento generalizzato dei diritti dei più deboli. È un grande segno di civiltà. I Paesi occidentali se ne erano già fatti carico, ma pensiamo a quanti altri Paesi hanno bisogno di questi stimoli, di questi pungoli da parte della comunità internazionale.

Convenzione a livello generalizzato di tutti gli altri Paesi rappresenterà, come il 1948 ha segnato per la Dichiarazione dei diritti umani, una soglia importantissima, una linea di demarcazione di ciò che era prima e di ciò che sarà dopo. come uscire da una specie di Medioevo statuale. Gli Stati si ammodernano, diventano Stati di diritto e, riconoscendo questo, si fanno sostanzialmente anche carico delle disparità esistenti all'interno degli stessi.

consentire ai disabili di partecipare alla vita della comunità con la massima indipendenza è proprio la realizzazione della democrazia in senso pieno

dovrà essere messa nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie opportunità. Infine, la partecipazione alla vita pubblica, sia politica che culturale, è un'innovazione di un peso enorme. Vorrei ricordare alcuni

rappresentato in quel momento dal ministro Paolo Ferrero, la Convenzione sui diritti delle persone disabili. Accanto alla firma del Governo italiano apposero la loro firma i due rappresentanti delle federazioni che raggruppano le associazioni delle persone disabili, la FISH e la FAND. Con grande enfasi la Convenzione - è stato qui richiamato - venne intitolata come la prima Carta universale dei diritti umani del nuovo millennio e, per le attese che essa ha suscitato nei Paesi sottoscrittori e tra le persone disabili e le loro famiglie, credo che tale sottolineatura abbia reso evidente una grande verità. Ci sono voluti dieci anni di dibattiti, incontri e raffinamenti successivi in cui i protagonisti non sono stati unicamente i rappresentanti degli Stati, ma soprattutto le persone disabili, le loro famiglie e le loro associazioni. In dieci anni è stato svolto un lavoro che appartiene ed onora il nostro Paese e che ha visto l'Italia tra le Nazioni che hanno sostenuto con forza le ragioni politiche, sociali ed umane che erano al fondamento della realizzazione di questo importante atto giuridico che vincola gli Stati a livello sovranazionale nella promozione e nell'avanzamento dei diritti delle persone più deboli e alle quali deve essere garantito il sostegno e la difesa dei propri diritti fondamentali. Il Governo Prodi si impegnò a ratificare entro il 2007 tale Convenzione. Purtroppo la fine prematura della legislatura non consentì di rispettare tale impegno, nonostante il 27 dicembre 2007 il disegno di legge contenente la ratifica stessa fosse stato approvato dal Consiglio dei ministri e inoltrato al Parlamento che non fece in tempo ad approvarlo in via definitiva. Il nostro partito ha ritenuto un dovere collettivo quello di mantenere fede a quell'impegno e all'inizio della legislatura la grande maggioranza del nostro Gruppo ha ripresentato il disegno di legge sollecitando così il Governo attuale a mantenere gli impegni presi nei confronti delle persone disabili. Oggi questo impegno viene portato a compimento in un ramo del Parlamento e ci auguriamo che possa presto diventare legge definitiva dello Stato. Siamo orgogliosi di quanto oggi sta avvenendo in quest'Aula, perché con questo provvedimento si riconoscono alle persone disabili dignità e diritti. Troppo spesso verso le persone più fragili ed indifese viene facile ricorrere al pietismo. Questa Convenzione cambia radicalmente il modo di affrontare il tema dei diritti e dell'uguaglianza delle opportunità per le persone svantaggiate: non atteggiamenti compassionevoli, ma dignità e tutele al passo con una società solidale ed accogliente per far vivere ad ognuno e al meglio la propria condizione, superando pregiudizi e stereotipi vecchi e ormai anacronistici. Quando mi sono occupata delle persone disabili, nella mia breve esperienza di Governo, ho tratto un grande insegnamento, vale a dire che il più delle volte disabili non si nasce. nel nostro Paese la disabilità dalla nascita è molto contenuta. Ma è durante l'arco della vita che incidenti, malattie, condizioni lavorative e sociali possono rendere improvvisamente una persona non più in grado di essere del tutto presente ed autosufficiente. L'allungamento della vita ci porta a convivere con malattie inedite e invalidanti, che riducono di molto la capacità di vita autonoma, e il peso per la famiglia e per chi ha il compito di accudire queste persone è notevole e grave. La disabilità è un mondo complesso. Quella fisica la si può affrontare e governare in modo più appropriato, mentre la disabilità psichica è devastante e molte volte conduce a tragedie umane e familiari perché spinge all'isolamento le famiglie e il disabile stesso. Ecco perché una legislazione compiuta e completa rappresenta un atto di civiltà parlamentare e giuridica, che onora la comunità internazionale ed il nostro Paese che l'ha sostenuta. Non ci convince lo strumento dell'Osservatorio previsto dal Governo, e lo abbiamo ampiamente argomentato. Vigileremo perché esso non sia un impedimento ed una sovrastruttura che rallenta il dispiegarsi delle potenzialità

dalla realizzazione del Fondo a sostegno delle persone non autosufficienti e non faremo mancare alle associazioni delle persone disabili il nostro appoggio e la nostra solidarietà. Per queste ragioni, ho il privilegio di annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

il Popolo della Libertà, per far fronte ad ogni forma di discriminazione ed esclusione dei disabili, si riconosce nella proposta di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, riconoscendosi nelle finalità della Convenzione di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, nella volontà di contribuire in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità. Donne, bambini e uomini dalle gravi povertà, colpiti altresì dal dramma della disabilità, trovino nell'attenzione dell'Osservatorio nazionale proposto gli strumenti contro ogni violazione della dignità della persona umana. Le misure legislative e amministrative, già presenti tra le vigenti norme dello Stato italiano, e le ulteriori che si adotteranno siano cogenti nell'impegno garantendo il superamento di logiche puramente assistenziali e sanitarie. Sono convinto che dalla sensibilità del Governo e dall'Osservatorio nasceranno iniziative formative e di informazione per un'adeguata sensibilizzazione in ogni ambito, da quello familiare a quello scolastico ed associazionistico, per accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità contro stereotipi, pregiudizi e pratiche dannose. Votiamo favorevolmente perché la disabilità, che è il risultato dell'interazione tra persone con menomazione e barriere comportamentali ed ambientali - come ci ha ricordato poc'anzi la senatrice Bassoli che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri, trovi nella forza espressa dal voto unanime del Parlamento la via del recupero, del reinserimento e della integrazione, eliminando emarginazione e favorendo inclusioni, creando premesse suggestive di reale partecipazione e tutela sociale. Siano norme forti contro i diritti negati per rompere il muro del silenzio, per non abituarci all'indifferenza. Occorre una naturale comprensione senza ricorrere ai giudici per garantirsi il diritto di una propria storia, di una vita libera, dove le disabilità non saranno più sbandierate come punti di forza. Oggi l'Italia ratifica una Convenzione ed istituisce uno strumento - l'Osservatorio che torna a far credere in un destino positivo chi delle difficoltà ha fatto la previsione ordinaria della propria vita.

a nominare, di concerto con il Presidente della Camera dei deputati, i due commissari mancanti, ponendo come termine le ore 24 di ieri. Sarebbe molto interessante sapere, non soltanto per tutti i senatori attenti o meno attenti alla questione, sia oggi che in passato, se in effetti la nomina d'ufficio è stata effettuata. Noi continueremo a ripetere fino alla alla noia, anche individuale, che siamo in patente violazione della legalità costituzionale in un contesto in cui si dovrebbero emanare regolamenti di partecipazione ad elezioni regionali prossime venture

di un argomento fondamentale, soprattutto perché stiamo discutendo la questione della sicurezza. Voglio ringraziare la Presidenza ed anche il Servizio dell'Assemblea e tutti i

«Il Tempo» per appellarsi ancora una volta al Governo del Brasile affinché Cesare Battisti ritorni. Tanti sono stati gli esponenti *bipartisan* che hanno aderito a questa grande iniziativa, che ha visto la partecipazione di esponenti di tutte le forze politiche. Voglio ricordare altresì l'intervento, oggi, di Olga D'Antona, parlamentare del Partito Democratico, che ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa. Sono qui per riconfermare l'essere un impegno anche del Parlamento italiano far sì che un assassino, responsabile di quattro omicidi condannato dalla giustizia italiana, possa ritornare e scontare nelle carceri italiane la pena che la magistratura gli ha assegnato.

mai messa all'ordine del giorno. Solo per curiosità chiedo ancora alla Presidenza di sapere se nell'ipotesi

anche a lei dico che informerò il presidente Schifani, però voglio ricordare che abbiamo avuto modo di discutere ampiamente le questioni economiche. Comunque riferirò. **Interrogazioni,